Signor Presidente, cari colleghi, lasciatemi iniziare questa mia relazione usando proprio la lingua dei segni, che

Oggi presentiamo infatti una norma di civiltà, provando a cancellare la vergogna di vivere nell'ultimo Paese in Europa, che non ha ancora una legge che riconosca pienamente i diritti essenziali delle persone sorde, in particolare di quelle segnanti. Lo dico in particolare a coloro che sentono più da vicino questa situazione - e sarebbe ora che anche in quest' Aula fosse possibile modo comprensibile per tutti coloro che hanno una disabilità uditiva, grazie ad un interprete LIS o ad una sottotitolazione - e che sanno bene cosa significhi non poter partecipare pienamente alla vita della propria comunità a causa dell'impossibilità di comunicare, per i quali le pari opportunità educative a scuola e all'università, ascoltare un telegiornale, spiegare ad un medico il malessere proprio o dei propri figli, ricevere informazioni in una stazione, ottenere un certificato da una pubblica amministrazione, far comprendere senza timore di essere fraintesi le proprie ragioni, davanti ad un giudice o ad un poliziotto, rischiano di essere ancora diritti negati. Inizio questa relazione dicendo che, con questo provvedimento il Senato, e spero presto anche la Camera dei deputati, alle persone con disabilità uditiva del Paese e provano ad abbattere una barriera che nega ancora a tanti, nel 2017, il pieno diritto di cittadinanza. Lasciatemi ripetere quest'ultima

nella discussione che faremo e che vorrei potessimo sviscerare e risolvere, per poterlo superare finalmente, dopo tanti e tanti anni; un dibattito che, se vogliamo, affonda le radici addirittura in un congresso che parlava di questi temi a Milano nel 1880. Sono davvero troppi anni e sarebbe bello che questo provvedimento riuscisse, tra le altre cose, a contribuire a superare una volta per tutte le divisioni del passato. Voglio dirlo con forza: il testo di cui stiamo discutendo non vuole dare ragione agli uni o agli altri, favorire qualche presunta *lobby* o un'associazione a discapito di un'altra. È finalizzato soltanto alla tutela delle persone sorde e non di uno o dell'altro operatore del settore. Insieme, in un lavoro molto bello di Commissione, abbiamo avuto l'ambizione di far fare un passo in avanti al nostro Paese nel più generale campo dell'inclusione di tutte le persone con disabilità auditiva, garantendo più diritti e cercando di ottenere più attenzione per chi convive con questo limite e posso dire che, grazie al contributo di tutti, credo si sia fatto davvero più di qualche passo avanti. Abbiamo ascoltato in questi mesi, anche attraverso decine di audizioni che ci hanno aiutato a capire bene e ad ascoltare davvero tutte le diverse posizioni - qualche volta anche a farle incontrare - le ragioni di ognuno: dagli esponenti della cosiddetta comunità segnante a quelli che difendono le buone ragioni dell'uso della lingua parlata e scritta per le persone sorde. Negli articoli di questo provvedimento non ci si è posto il problema di chi avesse più ragione fra oralisti e segnanti, anche se più e più volte questo ci veniva chiesto, ma credo che il compito del legislatore sia diverso: il compito del legislatore sia diverso: quello che abbiamo provato ad assolvere è di alzare il livello di tutela e di garanzia per tutti, sperando di aver contribuito così al superamento di antichi pregiudizi e di divisioni non più attuali e certamente poco utili alla causa delle persone sorde. Nell'ambito del principio, che abbiamo più e più volte ribadito, dell'assoluta ed inderogabile libertà di scelta da parte delle famiglie, senza dubbio questa norma introduce una novità che vuol essere un allargamento di opportunità. Come dicevo prima, dopo vent'anni una legge arriva al pieno riconoscimento della lingua italiana dei segni, o della lingua dei segni italiana, come è più giusto chiamarla, ed accanto a questa della LIS tattile, per le persone che hanno un'ulteriore difficoltà, le persone sordocieche. La LIS come strumento di piena cittadinanza, con la dignità di essere diventata negli anni vera e propria lingua, non semplice linguaggio, dotata di un suo specifico lessico, di una sintassi, di una grammatica, che permettono a chi la usa il medesimo livello di raffinatezza espressiva di una lingua parlata. Negli ultimi anni - è esperienza di molti - ci siamo fortunatamente abituati sempre più all'uso pubblico della LIS: alcuni, anche se troppo pochi telegiornali, il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, grandi eventi in cui sul palco compare il traduttore in lingua dei segni, la possibilità per gli studenti di usare questo strumento nelle università. E a testimonianza della ricchezza espressiva della LIS, sappiamo che sono sempre maggiori anche le occasioni in cui le persone sorde segnanti sono diventate protagoniste di eventi artistici legati alla poesia, al teatro, al cinema e ad altre arti espressive. fa dunque un primo grande passo, sottolineando la necessità di offrire servizi di qualità e di investire, ad esempio, sulla decisiva qualità degli interpreti, mettendo il nostro Paese al passo con la Convenzione delle Nazioni Unite che, parlando dei diritti delle persone con disabilità, approvava nell'Assemblea generale dell'ONU una dichiarazione del 2006 che riconosceva il ruolo della lingua dei segni «come forma di comunicazione, come mezzo di inclusione, come garanzia di libertà di accesso alle informazioni, come strumento di educazione, infine come espressione di identità culturale». Ma - è bene sottolinearlo proprio per cominciare a smussare e a smontare alcuni pregiudizi che ancora ci sono - fin dalla lettura del titolo appare chiaro che questo provvedimento non si limita al pur doveroso riconoscimento della lingua dei segni. Questa, anche perché elaborata nell'ambito della 1a Commissione, affari costituzionali, è una legge cornice, che punta ad allargare il campo dei diritti per il più pieno esercizio del diritto di cittadinanza da parte di tutti i sordi italiani, oralisti e segnanti. Una norma che ribadisce l'impegno della Repubblica ad utilizzare tutti i canali comunicativi e linguistici: la sottotitolazione, le nuove tecnologie, i servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, per eliminare tutte le barriere alla comprensione della comunicazione, per promuovere la piena inclusione scolastica ed universitaria, l'accessibilità ai luoghi di lavoro, alle strutture preposte alla salute, al patrimonio storico, artistico e culturale, ai trasporti, alle strutture ed ai servizi della pubblica amministrazione. Diciamolo con assoluta chiarezza: il richiamo alla LIS non è in alcun modo in contraddizione con la consapevolezza che il presente, e ancor più il futuro di chi nasce con ipoacusia, anche nelle forme di sordità profonde, è e dovrà essere sempre più quello di tendere alla padronanza della lingua scritta e parlata. Non mettiamo in contraddizione le due cose perché non lo sono. Se lo sono state in passato non è questo il tema che dobbiamo sottolineare. Ho avuto la fortuna di visitare in questi mesi strutture di eccellenza nel nostro Paese, in cui i bambini nati sordi profondi, per i quali vi era stata una diagnosi tempestiva, l'immediato utilizzo delle protesi, l'impianto di moderni dispositivi cocleari nei primissimi mesi di vita, si sono visti restituire dalla tecnologia e dalle cure di personale specializzato,

al recupero di una piena padronanza linguistica scritta e orale - si dice nel disegno di legge - deve tendere l'intervento di tutte le strutture pubbliche: da quelle sanitarie, chiamate ad attivare, attraverso lo *screening* neonatale, come richiamato nell'articolo 3, tempestivi interventi che evitino di consegnare nei primi decisivi mesi di vita i bambini a un isolamento che inciderebbe pesantemente sui futuri percorsi cognitivi; fino alle istituzioni scolastiche e universitarie, in cui si gioca, come sappiamo, la *chance* di piena cittadinanza di ciascuno di noi. Lasciatemi dire una parola in più proprio sull'investimento in formazione, cui sono dedicati gli articoli 5 e 6 in particolare. Il nostro Paese fa già molto in questo provvedimento si richiamano le tantissime azioni positive che già si esercitano in questo campo. L'Italia è stata pioniera nel superamento delle scuole speciali lo so anche per esperienza professionale; da pedagogista me ne sono occupato in maniera particolare - nell'integrazione dei bambini e ragazzi con disabilità nel gruppo classe, insieme a tutti gli altri coetanei normodotati. Ma l'esperienza di questi anni e le eccellenze che abbiamo incontrato, anche con il lavoro della Commissione - penso alla scuola di Cossato o all'istituto «Magarotto» di via Nomentana a Roma - ci dicono che forse è possibile fare ancora di più, e che i percorsi sperimentali di bilinguismo LIS-italiano, con l'ambizione di farli gemmare in almeno ogni Provincia italiana, possono garantire maggiormente la valorizzazione della diversità come reciproco arricchimento e concentrare su un numero limitato di classi risorse, innovazione didattica e collaborazione con la ricerca universitaria. Lasciatemi ricordare a questo proposito

Non era possibile intervenire in questo provvedimento per affrontarla, ma davvero auspichiamo che si possa quanto prima risolvere i problemi di una struttura che si è distinta per esperienza e competenza di assoluto livello, anche per i suoi dipendenti che in questo momento vivono una situazione difficile. Concludo riservandomi di ascoltare e di rispondere puntualmente agli interventi che in discussione generale sicuramente ci saranno e che spero ci aiutino a sviscerare fino in fondo i dubbi legati a questo a questo provvedimento, se ancora ce ne fossero. Faccio due ultime sottolineature che spero servano proprio a facilitare lo scioglimento di questi dubbi, anche perché mi auguro davvero che alla fine di questa discussione la votazione su un tema così sensibile sia ampia, trasversale, di tutto il Parlamento italiano, proprio perché l'attesa fuori da qui è molto grande. È un tema su cui credo la politica possa provare a non dividersi.

L'obiettivo che abbiamo perseguito è quello di allargare le opportunità, non certo di ridurle. Ed è evidente dalla lettura di ciascuno degli articoli del provvedimento. Ma lo voglio dire con ancora più precisione: chiunque pensi che riconoscere la LIS significhi imporla anche a chi ha scelto altri percorsi può davvero essere certo che non è così, non solo perché sarebbe contrario a questa norma e alla Costituzione, ma perché l'obiettivo del nostro lavoro va esattamente nella direzione opposta. Vogliamo che in futuro le nuove tecnologie permettano a tutti i bambini nati sordi in Italia di superare pienamente il loro *deficit*, e la legge va in questa direzione, ma crediamo sia giusto riconoscere che per decine di migliaia di persone adulte oggi la LIS sia uno strumento fondamentale di cittadinanza attiva e che studi scientifici italiani e internazionali confermano che il bilinguismo LIS-italiano può essere un valore aggiunto anche per i più giovani. Un ultimo riferimento all'articolo 15 ed al finanziamento di questo provvedimento. La stesura delle relazioni tecniche dei Ministeri ha permesso di ridurre di molto la previsione di spesa iniziale, ma penso sia importante sottolineare che i 2 milioni di euro, che probabilmente verranno individuati e allocati, saranno destinati alla copertura della previsione dell'articolo 3 relativa alla previsione ed alla diffusione dello *screening* neonatale nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) su tutto il territorio nazionale. Proprio lo *screening* neonatale, quello che abbiamo individuato come lo snodo decisivo per un precoce ed efficace percorso di acquisizione della lingua parlata e scritta oggi, purtroppo - ed è un'ulteriore vergogna - è un diritto accessibile solo a chi vive in quattro o cinque Regioni del nostro Paese; questa è forse la principale ingiustizia da superare e noi vorremmo farlo per dare piena attuazione alle previsioni di questa legge. Concludo con una citazione. Un autore che mi è caro, Elias Canetti, nel romanzo «La Lingua Salvata» racconta in modo mirabile modo mirabile quale sia il peso ed il condizionamento, positivo e negativo, delle lingue nella vita di ciascuno di noi: «Io credo infatti che faccia parte del sapere il volersi rendere manifesto e non contentarsi di un'esistenza nascosta». questa davvero l'ispirazione di questa legge e l'auspicio che ci regaliamo sperando di portare a compimento un provvedimento molto atteso al di fuori di questa Aula. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Puppato.

lo strumento che permetta al nostro Paese di vedere, da Sud a Nord, da Est a Ovest, la stessa attenzione da parte delle istituzioni pubbliche,

in relazione al fatto che oltre a queste realtà ne esiste un'altra che è stata inserita all'articolo 1 e di cui vado a trattare in particolare perché è da essa che è nato il mio interesse rispetto alla lingua dei segni. Al comma 3 dell'articolo 1 abbiamo previsto che le misure previste dalla presente legge si applichino in favore di persone con sola disabilità comunicativa non dovuta a sordità. Mi fa piacere leggervi una parte di una lettera

grazie ad essa si è inserita nella scuola primaria in modo assolutamente positivo. Il primo anno di scuola primaria per Lisa Fantin è stato un anno estremamente positivo. Cito un paio di frasi che questa mamma mi scrive e ne faccio dono a quest'Assemblea, per rendere comprensibile come la scuola italiana riesca contemporaneamente ad assumere quella evidenza di qualità eccellente, proprio per i rapporti umani che si creano e per la qualità didattica, ma, nel contempo riesca - ahinoi - a sprofondare nella difficoltà, se non nell'indifferenza, qualora cambino le persone e le istituzioni preposte. «L'*handicap* di mia figlia, la disprassia oro-facciale, la porta a non poter parlare. Non riesce a programmare il movimento della bocca e, quindi, ha difficoltà a fare uscire le parole a livello fonetico. Frequenta il primo anno della scuola «Pravato» di Paese. Ora siamo alla fine di quest'anno ed è stato - le devo dire - ricco di emozioni e di crescita per la bambina. Un ottimo lavoro da parte dell'*équipe* scolastica, sia per l'insegnante di sostegno che per quelle di ruolo nella classe. Il merito va a loro, per avere riconosciuto l'*handicap* di Lisa ma, contestualmente, aver permesso che ella fosse perfettamente inclusa». ma inclusa. Bene ha fatto, dunque, la Commissione sanità del Senato a insistere su questo tema rispetto alla normale e ordinaria integrazione. L'inclusione vera significa dialogo, significa quello che diceva adesso il senatore Russo, significa la possibilità di comprendersi, appunto, e di vivere contestualmente all'interno della società senza particolari problemi. Ebbene queste maestre hanno imparato da sole la lingua LIS per quello che era indispensabile, ma questa bimba ha avuto la fortuna di avere una insegnante di sostegno

Le ASL, la Provincia, la direzione scolastica non hanno voluto, o saputo, comprendere la difficoltà di questa famiglia nei di questa bimba, che tornava a casa da scuola ogni giorno più triste e più in difficoltà, con un rischio di danni neurologici e con un rischio davvero serio di demenza (siamo nei primi anni di vita, nell'ambito della costituzione di quella necessità di appartenenza al mondo che è così importante per esistere, come persone e come persone sociali). Ebbene, quel fatto stava avvenendo e i genitori, a questo punto, hanno deciso di spendere tantissimo per riuscire ad affiancare a questa bimba un insegnante, che loro stessi pagavano, e, nel contempo, ricorrere al TAR e costituire autonomamente dei corsi di formazione per gli insegnanti grazie all'aiuto dell'università di Venezia.

e la possibilità di esprimersi in una lingua conosciuta anche dagli altri. L'articolo 5, in questo senso, è un eccellente modello che ci mette finalmente al pari dei migliori Paesi europei. Concludo ricordando che, proprio all'interno di questo articolo 5, le amministrazioni pubbliche tutte competenti garantiscono la prestazione dei servizi volti al sostegno e all'inclusione di questi allievi, fornendo gli ausili tecnici e tecnologici, fornendo gli insegnanti di sostegno adeguati, gli assistenti alla comunicazione. Il MIUR si impegna a predisporre professionisti debitamente qualificati all'insegnamento della LIS e della LIS per i differenti ruoli di assistente alla comunicazione e di assistente all'autonomia, in modo da determinare *standard* nazionali nei percorsi formativi per l'accesso a tali professionalità. professionalità. Oggi è davvero un giorno speciale, perché inizia questo *iter* che permette, come diceva giustamente il relatore Francesco Russo, il diritto al rispetto e alla piena inclusione dei nostri bambini in questo Paese in tutti gli ambiti scolastici,

partecipazione ai problemi delle persone di cui ci occupiamo oggi. Mi permetto però di dire proprio a lei, signor relatore, che non dobbiamo vergognarci di essere italiani, né in generale e neanche su questo punto, perché, se è vero che fino ad oggi non c'è stata una legge specifica che riguarda i non udenti (i sordi), è dal 18 febbraio 1992 che c'è una legge che si occupa delle disabilità in generale.

Ci sono anche delle citazioni specifiche relative alla questione dei non udenti. Ad esempio all'articolo 9, viene specificamente citato il diritto delle persone non udenti a poter comunicare con la lingua dei segni. Pertanto, è bene fare dei passi avanti, ma non diciamo che l'Italia era indietro. L'Italia era avanti, perché la legge del 1992 è venuta prima di norme che sono arrivate a livello europeo e prima di norme che sono arrivate a livello delle Nazioni Unite; lasciamo stare poi le norme delle Nazioni Unite, perché in molti Paesi non c'è bisogno di avere delle minorazioni o delle disabilità per non poter usufruire neanche dei diritti fondamentali. Comunque, anche le nobili parole, spesso tali, delle Nazioni Unite sono venute dopo una legge concreta approvata in Italia, di cui non ha merito credo nessuno dei presenti, per questioni di anzianità. Per cui - ripeto - l'Italia non è indietro e non è un Paese incivile; non lo era allora e cerchiamo di fare in modo che non lo sia oggi.

la formulazione iniziale e quelle che si sono venute a creare durante i lavori in Commissione hanno suscitato notevoli preoccupazioni e prese di posizione, non da parte di di persone insensibili a questa problematica, ma proprio da parte di associazioni che riuniscono le famiglie o le persone

il Presidente della Società italiana di audiologia e foniatria e decine di professori di queste specialità la Federazione italiana per il superamento dell'*handicap*, che è stata anche audita in Commissione, le Famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi, l'Onlus Audientes, l'Associazione sordi e via

ricordiamoci che dobbiamo fare soprattutto un lavoro serio, che si attenga alla realtà, e sapere che anche con le migliori intenzioni si corre il rischio di fare qualcosa che vada al di là delle buone intenzioni, che non sempre può avere l'effetto desiderato. Ci sono - è bene che si sappia - varie alternative alla lingua dei segni. Chi usa e si trova bene con questo modo di comunicare deve essere supportato, e su questo non ci sono dubbi, ma sicuramente c'è concordia generale in quest'Assemblea. Non bisogna però tralasciare le altre tecniche, tra cui la lettura labiale,

e che si riferisce all'identificazione precoce della sordità e della sordocecità e agli strumenti atti ad attenuare e correggere i *deficit* uditivo e visivo.

Margaret Thatcher disse, facendo naturalmente discutere come spesso le accadeva, che nessuno si sarebbe ricordato - a cominciare da colui che ne narrò la storia - del buon samaritano se non avesse avuto i mezzi per provvedere al poveretto che era stato lasciato in un fosso pesto e moribondo.

o non siano sostenute dai mezzi approntati per metterle in atto o possano portare in direzioni diverse da quelle che noi tutti auspichiamo. Concludo il mio intervento sottolineando il pieno supporto del Gruppo di Forza Italia a politiche per il superamento di qualunque limite delle persone

Credo che uno dei capisaldi del disegno di legge sia proprio la libertà di scelta delle famiglie, che è la cosa più importante. Chi ha un problema di questo tipo da risolvere è giusto che

in grado di affrontare *handicap* di diverso tipo, ma sono privi di una specializzazione specifica. Credo che questa sia una questione su cui riflettere. È opportuno valorizzare quello che rimane della specializzazione in Italia, per consentire alle famiglie che lo vogliono, senza oneri, un recupero integrale del loro figlio naturalmente consentire il sostegno necessario, senza però dare particolari illusioni che nella scuola sia possibile recuperare con un'ora alla settimana il bambino in quelle condizioni. a un linguaggio dei gesti che naturalmente non sia in concorrenza con questi tipi di realtà, perché oggi un bambino è in grado di imparare sia a parlare sia ad apprendere la lingua dei segni e quindi - come ha detto il collega Malan

di cui apprezzo la relazione così compiuta, che finalmente davvero possiamo allinearci agli altri Paesi europei dando riconoscimento alla lingua dei segni italiana e alla LIS tattile. Ora finalmente siamo al pieno riconoscimento della lingua dei segni italiana. I provvedimenti legislativi che trovano una sintesi nel testo proposto dalla Commissione - sia chiaro - sono tutti indirizzati a una finalità: migliorare le condizioni d'inclusione nella vita sociale delle persone con disabilità uditiva o sordo-cieche nel processo di normalizzazione delle attività, nella facilitazione all'accesso all'istruzione, al mondo del lavoro e nel rapporto con la pubblica amministrazione. Tutti questi principi sono diritti sanciti nella Carta costituzionale e sono certo richiamati - come diceva poc'anzi il senatore Malan

Prezioso si rivela l'articolo 5 del disegno di legge per la garanzia della prestazione di tutti i servizi volti al sostegno e all'inclusione dell'alunno sordo con disabilità uditiva o sordo-cieco, tra cui la presenza, a seconda delle necessità di ciascuno, del docente di sostegno, dell'assistente alla comunicazione - nel caso di alunni sordi - e dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione - nel caso di alunni sordociechi dell'interprete in LIS e LIS tattile, di ausili tecnologici, di altre risorse e di operatori che assicurino la piena partecipazione e l'accessibilità alle attività scolastiche ed extrascolastiche. Devo dire che nella mia esperienza ho avuto ragazzi, studenti, ma anche assistenti amministrativi, nonché personale ATA sordo di cui ho seguito la difficile strada verso la normalizzazione.

che, in base alla libera scelta degli studenti sordi (libera appunto), purché su approcci scientificamente validati, con disabilità uditiva in genere e dei sordociechi e delle loro famiglie, promuovano il bilinguismo tra la lingua italiana parlata e scritta e la LIS o, nel caso di studenti sordociechi, la comunicazione totale. La Repubblica dunque promuove nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione l'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva, quali la LIS e la LIS tattile, e di ogni strumento tecnico e informatico accessibile e inclusivo idoneo a favorire la comunicazione delle, con le e tra le persone sorde e sordocieche, ivi inclusi *smartphone*, *tablet* e analoghi e analoghi dispositivi. Promuove altresì la prestazione di servizi d'interpretariato in LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire per tutte le persone sorde la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti alla generalità dei cittadini. Altri sono però gli articoli finalizzati a facilitare l'inclusione e a favorire l'accesso agli ambiti sanitari, al mondo della cultura, dell'arte e alla mobilità, attraverso mezzi di trasporto, e alla partecipazione politica. Al comma 2 dell'articolo 11 troviamo il disposto in base al quale la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, le Regioni e gli enti locali promuovono servizi d'interpretariato in LIS e LIS tattile e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento d'interesse generale. La modernità e la civiltà di uno Stato si misurano anche attraverso l'impiego diffuso delle tecnologie e un sistema di Stato sociale che garantisca pari diritti e il raggiungimento di un'uguaglianza e di una pari opportunità soprattutto per le persone che, loro malgrado, sono meno fortunate. Cito la convenzione ONU sul riconoscimento della LIS, che trova finalmente attuazione nel nostro ordinamento - sottolineo e ribadisco che siamo gli ultimi in Europa sia anche il preludio di un'estensione delle tutele garantite dalla legge n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, ovvero la possibilità di accedere a tutti i servizi all'interno degli ospedali, delle scuole e delle università. Al mondo della scuola e della formazione è noto come gestire le diversità sia un'operazione complessa, difficile e meritevole di andare avanti e fare ulteriori passi, come avverrà attraverso questa legge.

meritoria realizzata per raggiungere gli obiettivi che oggi sono qui davanti a noi e che mirano alla piena inclusione dalle più antiche scuole

Pagon e Thoman, raccolsero alcuni sordomuti di ambo i sessi per istruirli ed educarli con il metodo convenzionale. L'ispettore scolastico, un certo Valentino Stanig, apprezzati i risultati degli insegnanti, fondò lo Stabilimento per sordomuti che entrò a far parte dell'amministrazione pubblica nel 1840. Guardate cosa c'era e guardate cosa oggi non c'è. C'è sempre tempo, a volte, d'imparare dal passato.

meritevole soprattutto per quanto riguarda le disabilità plurime, cioè i sordociechi, e quanto sta facendo anche l'Istituto Regionale Rittmeyer di Trieste, scuola d'eccellenza nazionale e internazionale, le cui esperienze si sono rivelate preziose per favorire la piena partecipazione e inclusione sociale delle persone sorde e sordocieche alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana. Questo è fondamentale. In tutte le fasi, dalla culla alla fine della vita, viene garantito un diritto per chi non vede e non sente, che deve essere fatto valere seriamente ed efficacemente, eliminando le barriere della comunicazione e includendo sempre, con una comunicazione gestuale o tattile, tecnologica e soprattutto umana, chi vive nel silenzio e, a volte, nel silenzio e anche nel buio.

un argomento importante e interessante, che nasce dal desiderio di comprendere, analizzare e valutare la normativa ed eventualmente i progetti di bilinguismo per l'integrazione dei bambini sordi

la formazione degli schemi di adattamento, che assecondano la formazione e lo sviluppo della persona. Per questo motivo la costruzione dell'identità sorda per un bambino ha difficoltà a costituirsi, a integrarsi e a emergere nella società. L'isolamento sensoriale diventa isolamento comunicativo, con conseguenze dirompenti sul comportamento, quali l'irruenza, il disagio, l'instabilità, l'ansia, la paura e l'incomunicabilità.

ricordare che un bambino sordo ha le stesse potenzialità di apprendimento del bambino udente: la differenza tra i due bambini, di cui occorre tener conto nell'educazione, sta nell'uso privilegiato del canale sensoriale utilizzato nella comunicazione, che per i i bambini sordi hanno diritto di apprendere le due lingue: la lingua dei segni e la lingua italiana. La lingua dei segni italiana è una vera e propria lingua, con una sua grammatica e una sua cultura e, come tante, permette non solo di comunicare, ma anche di sviluppare il pensiero e le abilità cognitive. Occorre parlare dell'educazione bilingue del bambino sordo nella società italiana, considerando che la parola "sordità" viene generalmente utilizzata per indicare un *deficit* sensoriale uditivo: non un *handicap* fisico da mascherare e da curare, bensì una risorsa umana generatrice di cultura. Il problema della sordità ha le sue radici nel rapporto dell'individuo con la società: la sordità è invisibile e conoscibile solo al momento di comunicare. Così le persone sorde non sempre ricevono da parte degli udenti tutte le necessarie attenzioni e la disponibilità necessaria per comunicare e integrarsi. Questa esclusione causa un forte *stress*, soprattutto nei bambini, che aggrava notevolmente l'*handicap*. Tra le ragioni del comportamento aggressivo del bambino sordo c'è forse anche il senso di impotenza impotenza di fronte alla difficoltà di comunicare con i genitori, i compagni di scuola e gli insegnanti. Io stesso, signor Presidente, nel mio piccolo e a nome di tutto il Gruppo, ho presentato un

Abbiamo cercato di focalizzare l'attenzione soprattutto sulla disciplina dell'accessibilità alla comunicazione e dell'informazione nei luoghi pubblici e privati e sui rapporti con la pubblica amministrazione. Si è parlato anche di scuola, dove gli amministratori pubblici competenti garantivano la prestazione di tutti servizi per il sostegno all'integrazione degli studenti sordi, sordociechi e con disabilità auditiva.

Un'attenzione particolare si è avuta anche rispetto alla questione legata alle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo quali punti in cui è previsto un servizio di interpretariato in LIS.

non è un codice comunicativo universale, bensì esistono tante lingue dei segni quante sono le comunità sorde su tutto il pianeta, che - esattamente come le lingue vocali - sono nate spontaneamente. Le lingue dei segni sono molto diverse dalla gestualità che spontaneamente si utilizza durante una normale conversazione: a differenza dei gesti, infatti, esse sono un sistema di simboli relativamente arbitrari e di regole grammaticali che mutano nel tempo e che i membri di una comunità condividono

qual è il metodo più efficace nell'educazione al linguaggio del bambino sordo. Sono molte le variabili: il successo di un percorso di riabilitazione potrebbe dipendere dal metodo seguito, ma ogni bambino è unico ed è diverso. in particolare sull'uso dei metodi. Sono stati inventati e anche attualmente vengono proposti i più disparati metodi, ognuno dei quali veniva e viene considerato veniva e viene considerato spesso risolutivo. Fra questi metodi la contrapposizione più forte, per le diverse implicazioni educative, linguistiche, culturali e sociali, è stata quella tra il metodo orale e quello che, per semplicità, gestuale. Com'è noto, la lingua è forse il fenomeno più complesso che esiste e, quindi, la misurazione dello stesso è assolutamente difficile, se non obiettivamente impossibile. misurazione viene a essere applicata e richiesta su soggetti che hanno problemi di udito.

il relatore, che ha svolto un lavoro molto complesso e delicato nel portare a termine in Commissione il provvedimento in esame e voglio ringraziarlo per l'equilibrio con cui lo ha fatto, ma soprattutto per aver accolto gran parte delle indicazioni emerse dalla Commissione sanità, rispetto sia all'impostazione generale del testo, sia ad alcune specifiche questioni. Esprimo, quindi, un apprezzamento particolare per questo provvedimento che risponde a delle esigenze

C'è la visione di chi ritiene che le persone sorde debbano essere inquadrate come minoranza linguistica o come comunità di diversi: una posizione sostenuta da molti, anche da alcune associazioni. C'è, poi, un'altra posizione all'interno delle varie sfaccettature di altre visioni che ritiene, invece, che le persone sorde, anche nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, oltre che della nostra Costituzione, debbano essere considerate e tutelate nei loro diritti come persone, e non in quanto minoranze. ritengo che questa seconda visione debba prevalere, perché è sicuramente molto più inclusiva e molto più capace di dare risposte a tutti nel rispetto di quella libertà di scelta che giustamente è stata inserita nel testo. Penso che le persone sorde debbano essere rispettate come persone e non non in quanto minoranza linguistica. Per questo suggerirei di rivedere attentamente tutti i momenti in cui in questo disegno di legge si parla di bilinguismo, ovvero se sia il caso di fare riferimento al bilinguismo, di fatto riconoscendo la minoranza linguistica, o se non si tratti piuttosto di bisogni speciali delle persone. Trattarle come minoranze vuol dire riconoscere un'identità che rischia di separare anziché includere.

al fine di aumentare la reale possibilità di inclusione sociale - come giustamente si dice nel titolo del disegno di legge, opportunamente modificato - è necessario ribadire lo sviluppo di ogni forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, anziché focalizzare l'attenzione - come in qualche caso è rimasto nel provvedimento - solo sulla lingua dei segni e sulla lingua dei segni tattili. Sappiamo tutti anche grazie allo sviluppo tecnologico, esistono ormai modalità di comunicazione che possono facilitare e migliorare la possibilità di comunicazione delle persone sorde

ulteriormente sviluppate nel futuro, possano essere ricomprese nel provvedimento ed essere immediatamente applicate,

tutto quello che può essere fatto per prevenire le conseguenze di problemi uditivi, specie nei bambini, soprattutto alla nascita e ancora prima in gravidanza. E ringrazio per avere accolto il nostro suggerimento in tal senso. Anch'io ritengo, debbano essere messi a disposizione fondi per gli interventi sanitari. Sappiamo che, se diagnosticata precocemente o addirittura se si interviene durante la gravidanza della mamma, la sordità può essere affrontata molto più facilmente insegnando al bambino a parlare. Quando i bambini riescono a parlare nonostante i problemi di sordità - credo sia esperienza di molti di noi - è veramente il segno di una soluzione spettacolare:

diritti già sanciti da molte leggi, e qualche volta si è relativamente vaghi nel fare un'enunciazione. Penso, per esempio, all'articolo 14, che dà alle amministrazioni pubbliche la possibilità di monitorare e sanzionare senza dare ulteriori indicazioni, il che vuol dire, a mio

Mi domando allora, con grande attenzione e rispetto per tutte le posizioni, se costituire delle classi miste, con *curriculum* bilingue, lingua italiana e lingua dei segni, in cui le due lingue vengono insegnate a tutti gli studenti e in cui inevitabilmente saranno iscritti gli studenti sordi della scuola sia il modo migliore per socializzare e superare le difficoltà di questi studenti. So benissimo che ci sono esperienze positive al riguardo, la mia preoccupazione è che poi l'applicazione, non necessariamente, come quando è sperimentale, e solo in qualche caso viene fatta con la massima attenzione al rispetto delle persone che hanno più problemi degli altri e bisogni speciali, rischi di dare luogo a risultati che possono non essere i migliori. La mia preoccupazione è che si pensi che possano esserci classi bilingue in cui alla lingua italiana si affianca la lingua dei segni, che vuol dire riconoscere

in molti casi si parla di promuovere giuste azioni e strumenti che devono essere adottati a sostegno di queste persone, in altri casi si parla di garantire. Se si dice garantire, bisogna metterci i soldi e bisogna essere capaci di dare un'attuazione effettiva; se non si mettono i soldi, scriviamo promuovere.

Salutiamo la dottoressa Shoshanna Makover, capo Ufficio resoconti, il dottor Yitzchak Yehuda, direttore progetti applicativi, e il dottor Oren Bar, direttore del settore ricerca e sviluppo

Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, debbo anzitutto esprimere la mia soddisfazione perché, soprattutto negli ultimi mesi, quest'Aula si è trovata più volte ad affrontare le tematiche legate alla disabilità. Penso al dibattito di martedì sulle persone affette da disabilità intellettiva e da sindrome di Down, ma penso soprattutto a una legge di grande civiltà quale il dopo di noi. Nelle scorse settimane ho personalmente preso parte a diverse iniziative sul mio territorio, come l'assemblea di ANFFAS, quella dell'Unione ciechi, l'inaugurazione della nuova sede della sezione di Trento dell'Ente nazionale sordi. Li menziono tutti, per dire come in ciascuna di queste circostanze ho potuto apprezzare i tanti passi in avanti che sono stati compiuti per garantire una migliore qualità della vita, una migliore forma assistenziale ai disabili e alle loro famiglie, ma soprattutto per aumentare il grado di accesso alla vita comunitaria. Certo, come abbiamo ribadito anche durante la seduta dell'altro ieri, c'è ancora tanto da fare per rimuovere tutte le barriere materiali e culturali che ancora esistono. In Italia siamo spesso all'avanguardia per quanto riguarda i principi e le enunciazioni, ma troppo spesso siamo carenti sul piano dell'attuazione dei diritti. La lingua dei segni per sordi, sordociechi e disabili uditivi è una vera e propria lingua, con una propria specifica morfologia, sintattica e lessicale, e non solo una modalità d'espressione della lingua parlata. Ne esistono più di trenta riconosciute al mondo ed oggi, come ha detto bene il relatore Russo, siamo l'unico Paese europeo, assieme al Lussemburgo, che ancora non ha riconosciuto la lingua dei segni dopo la Convenzione ONU di New York del 2006, che è stata poi ratificata dal nostro Paese nel 2009. Il riconoscimento della lingua è essenziale per garantire a tutti il pieno accesso al sacrosanto diritto di potersi esprimere nella propria lingua e, quindi, è un tema non molto diverso da quello di tutte le minoranze linguistiche. Sappiamo bene che non si tratta solo di un fatto simbolico, ma che si tratta di un diritto sostanziale, che non può più essere rimandato nel tempo: in televisione come nei grandi eventi pubblici l'interprete LIS è sempre più presente, a riprova di una sensibilità sociale cresciuta nel tempo, cui adesso anche le istituzioni devono adeguarsi, colmando il colmando il ritardo che si è venuto a creare. Il provvedimento che oggi discutiamo ha avuto un percorso articolato ed è assolutamente positivo che si sia giunti a un testo unico, a dimostrazione che questo è un tema su cui le forze politiche devono trovare la convergenza. Molto importante è stato il lavoro fatto in Commissione e credo vada dato atto a tutti i suoi componenti, ai presentatori delle proposte di legge, al relatore, a tutte le colleghe e i colleghi che hanno lavorato sul provvedimento. È stato un lavoro di grande impegno, che ha coinvolto molte associazioni e realtà operanti nel settore e che ne ha raccolto le testimonianze, le richieste e il prezioso contributo d'esperienza. Voglio ringraziare in particolare l'Ente nazionale sordi e tutte le altre realtà che hanno collaborato e che garantiscono sul territorio la possibilità per tutte queste persone di condurre una vita più accettabile. Non ho dubbio nel dire che senza di loro, senza queste realtà preparate e motivate, oggi la nostra società potrebbe garantire ben poco. Il risultato di questo lavoro è nella completezza del provvedimento, che affronta davvero una pluralità di questioni, tutte importanti. Per ragioni di tempo vado per titoli: la prevenzione e l'identificazione precoce di fenomeni di sordità, gli interventi di sostegno psicologico, la costituzione di centri specializzati, l'aumento dell'accessibilità attraverso le nuove tecnologie e lo sviluppo di *software* dedicati; l'accessibilità universale agli ambienti, agli edifici, alle istituzioni e agli eventi artistici e culturali; le campagne di sensibilizzazione pubblicitaria; l'accesso ai servizi di emergenza e pronto intervento e alla pubblica amministrazione; la disponibilità di servizi di interpretariato e i corsi di formazione per gli interpreti; la disponibilità di insegnanti di sostegno e assistenti di comunicazione nelle scuole; l'accesso all'istruzione universitaria e postuniversitaria; l'accesso ai trasporti pubblici. Il mio auspicio è che, una volta approvato il testo, si faccia in fretta con i decreti attuativi, ma soprattutto che, al di là di quelle stanziate, si trovino tutte le risorse indispensabili per garantire effettivamente un diritto che è sacrosanto ed è sancito dalla Costituzione. Per troppi anni alle persone affette da disabilità uditiva è stato negato il pieno diritto di cittadinanza. Con questo provvedimento, che ha illustrato molto bene il relatore, viene finalmente ribadita la libera scelta da parte della famiglia. È una scelta di civiltà e mi auguro che nei prossimi mesi l'Italia non sarà più il fanalino di coda dell'Europa. Lo dobbiamo a tutti coloro che vivono questo stato di grande difficoltà e di grande disagio. Certo, viene prima la cura e si sono ottenuti grandi risultati nel campo della medicina; io stesso li ho potuti verificare e per questo dobbiamo continuare ad investire anche nella ricerca. Oggi, però, compiamo un primo passo importante, che risponde a una battaglia di civiltà che migliaia di persone e di famiglie stanno portando avanti da anni. È iscritto a parlare il senatore Lepri. Ne ha facoltà.

inclusione dei ragazzi sordomuti o sordociechi determinò - non credo di sbagliarmi - in non pochi casi anche degli errori e dei drammi.

ha sempre sorpreso il fatto di incontrare tante persone avanti negli anni che, avendo frequentato queste scuole specializzate, che nel frattempo erano state chiuse, erano tutte capaci di parlare e in non pochi casi anche di intendere quello che noi rappresentavamo loro, pur essendo pienamente pienamente e totalmente non udenti. Allo stesso modo, sorprendeva, non piacevolmente, vedere tante persone giovani o di mezza età, successive alla chiusura di quelle scuole, non essere in grado di proferire parola e parlare solamente

ho sempre combattuto l'istituzionalizzazione e la segregazione di persone con qualche forma di difficoltà o di *handicap*. Tuttavia, la questione andava e va affrontata oltre gli steccati ideologici che hanno caratterizzato il dibattito degli ultimi anni ed è per questo che mi pare molto felice la sintesi che è stata fatta dal relatore e da chi ha collaborato con lui, perché in realtà non c'è un'alternativa tra la volontà di inclusione nella normalità e l'esigenza di interventi specializzati. quindi benissimo ciò che in non pochi casi viene detto: inserimento in contesti di normalità; impianti quando servono; prevenzione; strumenti tecnologici; *screening* neonatale; diagnosi precoce. Tutto ciò è assolutamente fondamentale. Non possiamo evidentemente pensare che la comunità delle persone sorde debba essere messa in un recinto e

di normalità, con insegnanti specializzati di sostegno, sapendo che comunque è molto difficile che la sola attività di sostegno in un contesto di normalità possa consentire consentire al bambino e al ragazzo di acquisire la capacità di parlare e di intendere. Vanno bene anche le classi miste e ogni sperimentazione che possa favorire forme favorire forme didattiche diverse, ma anche - lo sottolineo - la promozione della lingua dei segni e la sua diffusione nelle diverse forme: tattili, tecnologiche, per sottotitolazione,

combattersi in nome della comune difesa e promozione dei bambini, dei ragazzi e dell'intera comunità dei sordi. Ora dobbiamo guardare avanti e credo che questo provvedimento compia un passo davvero decisivo. Mi auguro che il Parlamento

perpetuare questa tradizione e questo orgoglio italiano, sia pur con ritardo, per promuovere davvero la vita delle persone e delle comunità sorde.

intelligentemente richiamato l'Assemblea agli aspetti più concreti di un vissuto che alcune volte, nel merito della disabilità

a obiettivi di inclusione, di socializzazione e di rispetto dei diritti individuali, oltre che di mitigazione della diversità. Questi sono i capisaldi del disegno

la soddisfazione espressa negli interventi fin qui succedutisi trovi giustificazione nel sapere che forte sarà l'impatto,

le disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, si compie un importante passo in avanti per realizzare una sempre maggiore inclusione sociale di quel mondo fatto di persone che

«le informazioni fornite prima del *test* dovrebbero offrire al potenziale utente la possibilità di comprendere ciò che gli viene comunicato e di esprimere le proprie valutazioni e le preoccupazioni relativamente ai vari aspetti del *test* Nel caso delle persone non udenti deve essere presente al colloquio un interprete della lingua dei segni, ed è utile avvalersi anche dell'ausilio di materiali scritti Questo provvedimento sarà utile al disbrigo di ogni altro atto, sia esso di natura pubblica o privata per il quale la legge abbia previsto che il contraente, muto o sordomuto, sia assistito da un interprete di fiducia atto a comunicare con lui attraverso la lingua dei segni o mezzi convenzionali,

perché naturalmente facilita l'intenzione di allargare le possibilità di applicazione della lingua dei segni ad un maggior numero di trasmissioni oltre ai telegiornali.

L'articolo 3 della nostra Costituzione proclama la pari dignità sociale e l'uguaglianza di tutti i cittadini. Oggi l'Italia, in questo ramo del Parlamento, intende tagliare un traguardo che si può certamente definire storico, adeguandosi al resto dell'Europa con il riconoscimento della lingua italiana dei segni per la tutela e la promozione dei diritti delle persone non udenti. Come dicevo, l'Italia si adegua all'Europa, dove la LIS ha avuto un riconoscimento al più alto livello con due risoluzioni del Parlamento europeo,

Cari colleghi, quando parliamo di persone non udenti e, più in generale, di persone con disabilità, proprio per applicare concretamente nella nostra legislazione il principio enunciato nell'articolo 3 della Costituzione, diventa indispensabile superare le barriere, a tutti i livelli, non solo quelle fisiche, ma anche e soprattutto quelle sociali, culturali e, in questo caso, anche linguistiche. Questa è la battaglia che, da anni, ci vede impegnati, insieme al mondo dell'associazionismo dei sordi, per il riconoscimento della LIS. Si tratta di uno strumento che consente, in primo luogo, ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo nell'ambito della propria comunità.

Una volta che verrà riconosciuta la lingua dei segni, dunque, bisognerà assicurare l'accesso all'istruzione per mezzo di questo linguaggio. Capite bene, pertanto, quanto sia importante oggi

italiano con la legge n. 18 del 2009 per tutelare espressamente la specificità delle persone sorde, in Europa solo Italia e Lussemburgo non hanno proceduto al riconoscimento della LIS. Questo riconoscimento è un grande segno di civiltà; si tratta di un'iniziativa senza bandiere politiche perché ha a cuore gli interessi delle persone. Difatti, questi lavori non hanno colori di appartenenza, ma valori di appartenenza. Con il riconoscimento della LIS, le barriere della comunicazione possono essere abbattute, favorendo l'integrazione tra mondo dei sordi e mondo degli udenti. Ricordo uno dei tanti progetti che negli anni è stato fatto e che è venuto a mancare, rispetto al

il diritto ad ogni persona sorda di scegliere come comunicare e integrarsi nella società, garantiamo realmente l'accesso all'istruzione, alla cultura, alla comunicazione, all'informazione, a una vita sociale oltre che lavorativa. Così abbatteremo un «muro» che oggi divide la nostra società e, al contrario, costruiremo un «ponte» verso l'eguaglianza per garantire la pari dignità sociale e l'eguaglianza di tutti i cittadini. Forse

un obiettivo fondamentale: riconosciamo formalmente, anche in Italia, la LIS. Credo che questo sia un provvedimento che oggi non possiamo permetterci di non votare e di non far votare a questa Assemblea. Per questo, vi ringrazio dell'attenzione.

pudore, se non imbarazzo, che prendo la parola su questo argomento, ringraziando il relatore per gli sforzi profusi nell'intento di trovare soluzioni a problemi molto complessi. Pudore e imbarazzo in ragione dal fatto che per me l'approfondimento di questo tema è cominciato venticinque anni fa, nel corridoio di uno dei più noti nosocomi italiani quando, uscendo dalla sala per i potenziali evocati, un giovane dottore, forse con eccessiva fretta, a sua volta per nascondere un grande pudore e un grande dolore, rivolgendosi a mia moglie e a me

questo perché credo che la sollecitazione venuta dalla collega Dirindin, la quale ha chiesto in modo inequivocabile di distinguere tra il disporre, da parte dello Stato, diritti diritti ordinati a un principio che si riconosce nella persona in quanto tale e non nella persona perché le si attribuisca una privazione di essere, cioè una mancanza, un problema, principio ribadito anche nell'intervento del collega Lepri, debba essere l'elemento realmente dirimente perché possiamo elaborare una buona legge.

in ordine a qualcosa che non si è fatto negli anni precedenti e che troviamo agevole e ottimo fare in questa circostanza, ma soprattutto si propone come piattaforma giuridica per i diritti di cittadinanza di tutte le persone sorde, di tutte le persone con disabilità uditiva. Perché lo sia, allora, se è legge quadro, deve avere una denominazione che tenga conto non solo dei problemi di tutti, ma anche di ciò che quei tutti immaginano come l'approccio più conveniente, più utile e più ragionevole per la soluzione dei problemi. Voglio essere molto concreto: il relatore Russo ha detto che stiamo superando un problema e un ritardo;

che valorizza strumenti tecnologici e che ci porta più avanti nel tempo, perché con l'aiuto della tecnologia troviamo risposte adeguate a problemi che vengono da un tempo lontano e che tanto hanno segnato nel dolore i doveri e i diritti di una generazione. generazione. Questa rivoluzione tecnologica ha segnato anche il mondo della sordità e della disabilità uditiva e va tenuta in conto da parte dello Stato, proprio perché lo Stato è garante e non padrone della vita della gente. E proprio per essere uno Stato garante, si sforza di comprendere l'approccio di quei molti che oggi nel dibattito devono poter vedere riconosciuta la propria voce. Un gruppo di ragazzi minorenni, che vanno ancora a scuola

signor Ministro della salute, signor Ministro della cultura, ciò che segue è una richiesta da parte dei sordi italiani che vogliono parlare la loro, la vostra, la nostra lingua, ovvero l'italiano e non condividono alcuni passi chiave della legge attualmente in discussione in Parlamento circa il riconoscimento della lingua dei segni italiana». Non ho letto questo *incipit* per creare un elemento di divisione di legge in discussione vuole avere l'ambizione descritta dal collega Russo, deve essere capace di essere piattaforma utile dal punto di vista giuridico nell'interesse dei diritti di tutti. Chiedo allora, con molta semplicità, al collega Russo: perché non diamo a questo strumento normativo la denominazione di «legge quadro per il riconoscimento e la promozione dei diritti di cittadinanza di coloro che hanno disabilità uditiva»? è che semplicemente non faremo un adeguamento semantico per venire incontro anche agli altri sordi, ma ci vieteremo di comprendere che il male è privazione d'essere. Chi di noi penserebbe di trovare risposta al problema di coloro a cui mancano una o due gambe incitando a non fare le protesi? E allora, proprio perché dobbiamo riconoscere che sul tema della sordità c'è un problema di culture che si compongono e possono comporsi in modo diverso, non possiamo, come legislatori e come Stato, non far sentire la nostra preoccupazione concreta e la nostra capacità reale di rispondere a un bisogno senza stravolgere il senso fondamentale di ciò che la collega Dirindin ha detto: vale a dire che le persone si aiutano in quanto persone, che le persone hanno e maturano diritti in quanto tali e che il riconoscimento dei diritti della persona precede e non preclude mai la possibilità di andare incontro alle specifiche richieste e agli specifici possibili bisogni. Solo questo chiedo e lo chiedo, lo ripeto ancora, con pudore e con imbarazzo, non voglio che nessuno dei momenti vissuti nella solitudine, nella fatica e nella fragilità in questi venticinque anni possa rappresentare il modo con cui cerco di definire e chiudere le istanze e i problemi e il modo appassionato con cui chi l'ha vista diversamente da me ha cercato di stare vicino al diritto dei propri figlioli. Questo chiedo al relatore e alle forze politiche, soprattutto perché quella prospettiva di novità, il modo cioè in cui vogliamo dire che l'Italia, che era indietro su questo punto, ora potrà stare più avanti, deve saper leggere esattamente quello che in tutti questi anni è avvenuto. Per me è stata un'esperienza molto concreta. Fino a Fino a qualche anno fa, come ricorderanno molti colleghi, l'esperienza dell'impianto cocleare era preclusa dal più semplice dei problemi: nel prontuario sanitario nazionale quel passaggio era indicato come intervento di chirurgia estetica. C'è voluto un Ministro di quella parte dello schieramento, Umberto Veronesi, che in pochi minuti, ponendosi il problema con molto pragmatismo, ragionevolezza e semplicità lo ha risolto aprendo nuove prospettive nel campo dei diritti a molti sordi italiani.

Solo il Lussemburgo ci fa compagnia in questo ennesimo *record* negativo, mentre Austria, Finlandia e Portogallo hanno addirittura inserito la lingua dei segni in Costituzione. Pensate quanto sono avanti! legge in esame è più che mai urgente, poiché i soggetti affetti da problematiche e disagi strettamente legati alla vista e all'udito sono nel nostro Paese circa 189.000, dato che peraltro, secondo l'ISTAT, è in costante crescita.

visto che su una popolazione disabile di 234.788 ragazzi, anch'essa in costante crescita, risultano addirittura essere 9.885 i bambini e i ragazzi con disabilità sensoriali legate alla vista o all'udito, condizione che nel 38,1 per cento dei casi si associa a disabilità intellettiva, cento a disabilità di tipo motorio e nel 20 per cento a disturbi dello sviluppo e del linguaggio, mentre il 40 per cento dei bambini, soprattutto quelli con disabilità visiva, ha gravi problemi nell'apprendimento. Il testo che stiamo discutendo intende introdurre l'insegnamento della LIS nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e nelle università; prevedere l'utilizzo di nuove tecnologie per la sottotitolazione nelle trasmissioni televisive; inserire gli interventi diagnostici per l'individuazione precoce delle disabilità uditive e visive tra i minori nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni, al fine di poter ottimamente calibrare i necessari interventi protesici e logopedici; promuovere la ricerca scientifica e tecnologica per favorire un maggior impiego delle tecnologie visive

sia come singolo individuo che come soggetto appartenente a una comunità più ampia. Questo è quanto prevede il disegno di legge al nostro esame. Un traguardo, l'approvazione di questo atto, al quale però fa da contraltare la grave crisi economica di alcuni degli istituti statali per sordi presenti sul territorio nazionale. Cito, su tutti, quella in cui versa l'Istituto statale per sordi di Roma, che rischia l'imminente chiusura se non si procederà al recupero dei finanziamenti mai erogati all'istituto negli anni precedenti, quantificati in circa 19 milioni di euro, nonché all'assegnazione di un contributo economico annuo in attesa che venga rapidamente ultimata la sua trasformazione in ente nazionale. Con questa chiusura sarebbero a rischio molte delle attività di assistenza e supporto, ma anche di formazione, garantite dall'istituto in questi anni, peraltro richiamate nel disegno di legge dall'aggiornamento professionale degli operatori LIS all'attività di ricerca nell'ambito delle problematiche delle persone sorde, passando per il sostegno alle scuole e alla formazione degli insegnanti. Anche in questo caso occorre l'impegno di tutti, per far sì che le norme di civiltà contenute in questo provvedimento non rimangano lettera morta. La scuola su queste tematiche ha un ruolo fondamentale. Voglio soffermarmi sull'articolo 5 del disegno di legge, riguardante l'inclusione scolastica, che conferisce al il compito di garantire agli studenti sordi, sordociechi o con disabilità uditiva in genere, l'apprendimento della LIS e della LIS tattile o di ogni altra forma comunicativa efficace per la loro inclusione. Inoltre, sempre nello stesso articolo, viene riconosciuta al MIUR la prerogativa di definire i requisiti formativi che devono possedere i docenti che si occuperanno dell'insegnamento della LIS e della LIS tattile o del sostegno

in molte realtà territoriali addirittura drammatica, con molte cattedre di sostegno che risultano ancora vacanti, con il diritto allo studio, sancito dall'articolo 34 della nostra Costituzione, che viene continuamente violato che voi continuamente violate! - e con le famiglie che si trovano smarrite, quasi abbandonate, incapaci di affrontare situazioni di questo tipo, anche per l'assenza all'interno degli istituti scolastici di una figura professionale di riferimento, che faccia da raccordo con il minore e consenta a quest'ultimo di superare brillantemente i disagi e le difficoltà che caratterizzano e influenzano le varie fasi del suo percorso di crescita. Su quest'ultimo aspetto è condivisibile la previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge, secondo cui «La Repubblica promuove (...) interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le rispettive famiglie, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o sordocecità», perché si inserisce nel solco di un personale e costante confronto con studiosi e esperti del settore sul tema del ripristino della figura professionale del pedagogista all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, soprattutto per la prevenzione di situazioni critiche e disagi vissuti da bambini e ragazzi, anche riconducibili ad aspetti relazionali, emotivi e affettivi. Mi auguro che il nostro impegno non si esaurisca qui, ma soprattutto mi auguro che il vostro impegno non sia la solita marchetta elettorale e che l'*iter* di approvazione del disegno di legge abbia un'accelerazione alla Camera dei deputati. A quanto vedo, però, già questa mattina

il testo del disegno di legge sul riconoscimento della lingua italiana dei segni oggi all'esame dell'Assemblea è il frutto di un lungo lavoro svolto dal relatore Francesco Russo e dai colleghi della Commissione affari costituzionali, che ringrazio

i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione. Dopo diversi anni di attesa, i contenuti di tali previsioni prendono finalmente forma nel testo che oggi esaminiamo, in un processo lungo e faticoso. Come ricordato anche dal senatore De Poli De Poli e dal relatore, l'*iter* è partito dall'esame di ben cinque disegni di legge, poi confluiti in un unico testo, che avevano come principale obiettivo quello di giungere al riconoscimento della lingua dei segni (LIS) e di favorirne l'utilizzo pressoché in tutti gli ambiti, dalla scuola all'università, dai *mass media* al mondo del lavoro, dagli organi giurisdizionali alle strutture sanitarie. Tra di essi, c'è anche quello a mia prima firma, sottoscritto da molti colleghi, l'atto Senato n. 1019, presentato nell'agosto del 2013, prevedeva tra l'altro il riconoscimento della LIS allo scopo di consentire e agevolare il suo utilizzo nei procedimenti giudiziari, civili e penali, e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni e con gli enti locali. L'esame in L'esame in Commissione è durato oltre due anni ed è stato caratterizzato dall'audizione di esperti, associazioni, interpreti ed altri soggetti competenti in materia, che hanno fornito le proprie considerazioni ed osservazioni al fine di migliorare ed arricchire il testo presentato dal relatore. L'obiettivo di questo provvedimento è di riconoscere e garantire i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva. da poco, che in Italia le persone sordocieche sono 189.000. Sono in una situazione di grave solitudine e spesso di completa dipendenza dagli altri e di queste 108.000 sono praticamente confinate in casa, non essendo in grado di provvedere autonomamente a sé stesse, anche perché hanno altre disabilità. Sappiamo anche che circa 20.000 persone assommano

queste diventino poche perché saranno autonome. Questo è l'obiettivo del provvedimento: l'autonomia e i diritti di tutti. Proprio per riconoscere i loro diritti costituzionali, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento, la Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati

le indagini preventive in gravidanza, lo *screening* neonatale, la diagnosi audiologica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce abilitativo e riabilitativo, perché solo attraverso la diagnosi precoce abbiamo la possibilità di intervenire tempestivamente attraverso le protesi. È bene ricordare che le misure previste in questo articolo si applicano su tutto il territorio nazionale - bene ha detto il nostro relatore - in quanto considerate come livelli essenziali delle prestazionali, ai sensi della Costituzione. Con il secondo pilastro si specifica che il riconoscimento della lingua dei segni si realizza nell'ottica del del bilinguismo, conferendo alle famiglie la possibilità di utilizzare anche - e sottolineo «anche» - questo strumento per il proprio figlio affetto da ipoacusia o sordità. È una possibilità, una facoltà, ma non certo un obbligo: chi predilige l'approccio oralista non sarà mai proprio mai - obbligato a imparare la lingua dei segni e men che meno sarà costretto a farne uso a scuola o in altri contesti sociali. La libertà di scelta è un caposaldo e un diritto a non essere discriminati, ed è fondamentale in questo disegno di legge (articolo 2). quando una famiglia decida di ricorrere alla lingua dei segni, grazie a questa norma dell'ordinamento italiano, è garantito l'insegnamento di questa lingua nei percorsi formativi ed educativi, attraverso la presenza a scuola dell'assistente alla comunicazione, dell'interprete oltre all'insegnante di sostegno. Si garantisce, quindi, l'accesso a modelli educativi su libera scelta. In quest'ottica, il riconoscimento della LIS diviene strumento che l'ordinamento predispone per la tutela dei diritti delle persone sorde. Per quanto riguarda l'inclusione scolastica, si promuove l'attivazione di classi miste di studenti udenti e sordi con un *curriculum* bilingue. Noi abbiamo un esempio virtuoso, quello della scuola di Cossato, dove, dal 1994, c'è un progetto nato come sperimentale che, però, dura da ventitre anni: lì, dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado, attraverso la primaria, si forma un gruppo di alunni sordi che acquisisce la LIS come lingua naturale, insieme ad alunni udenti come lingua naturale, insieme ad alunni udenti che impiegano la LIS come seconda lingua il più precocemente possibile. L'esperienza maturata da questo progetto dimostra come l'intervento linguistico su bambini sordi, che poi prosegue nelle scuole superiori, è efficace proprio se iniziato quando sono piccoli, perché il bilinguismo favorisce l'inclusione degli alunni sordi che, comunicando in due lingue diverse, hanno la possibilità di un completo scambio di conoscenze. Abbiamo anche delle verifiche su questo, i monitoraggi fatti dal CNR, la collaborazione con l'università di Milano-Bicocca e con la «Ca' Foscari»; progetti con numerosi convegni nazionali e internazionali cui la scuola ha partecipato, con università straniere che vengono a studiare questo modello. Vi do anche dei numeri: diversi dati ci dicono che quattro ragazzi si sono già laureati, uno deve discutere la tesi a breve, tre sono iscritti all'università, sette hanno concluso gli studi delle scuole superiori, sei stanno frequentando la scuola superiore con grande successo. Sono risultati davvero rilevanti. Il MIUR è chiamato, poi, a definire, sentito un tavolo di esperti, gli *standard* nazionali dei percorsi formativi per l'accesso a queste professionalità che servono all'interno dei suddetti percorsi. Vorrei evidenziare un ordine del giorno, che ho presentato per l'esame in Assemblea, per chiedere la revisione dei criteri previsti dalla legge n. 107 del 2010 per il riconoscimento della sordocecità, garantendo alle persone sordocieche pieni diritti, oltre all'accesso alle specifiche previsioni normative disposte. L'attuale definizione di sordocecità, infatti, ha comportato l'esclusione formale di un numero considerevole di persone (ricordavo 189.000) che, pur presentando contemporaneamente una disabilità visiva e uditiva, hanno perso l'udito dopo il compimento del dodicesimo anno di età. Non è, dunque, agli effetti di legge, considerato

affermando ancora una volta che la vita delle persone sorde, sordo cieche e con disabilità uditiva più o meno grave fa i conti ogni giorno con le invisibili barriere della comunicazione e della relazione. Nel testo unificato si prendono in considerazione tutte le diverse esperienze di vita, le scelte familiari e la complessità della sordità, affermando innanzitutto il principio della libertà di scelta, il principio di trovarsi all'interno di una comunità educante, che si interessa, che cura le persone, ma soprattutto ha cura del percorso di crescita dei nostri bambini e dei nostri alunni. Le persone sorde e le loro famiglie hanno il diritto di scegliere la modalità di comunicazione e di accesso alle informazioni che prediligono, nel pieno rispetto della loro autonomia e della loro integrità personale.

ha partecipato apportando il proprio contributo sanitario e scientifico, anche in materia di cooperazione internazionale, per la prevenzione e il contrasto a malattie ed epidemie. Ad oggi sappiamo che parteciperanno a tale Assemblea 194 Stati, ma Taiwan

di una situazione che denunciamo contraria allo spirito e alle finalità dell'Assemblea mondiale della sanità e dell'Organizzazione mondiale della sanità che, nel loro atto costitutivo, nel loro statuto, stabiliscono di operare al di fuori e al di sopra di ogni motivazione razziale, religiosa, politica ed economica, perché il loro solo obiettivo è quello di tutelare la salute del genere umano. Virus, malattie ed epidemie non finiscono con i confini nazionali, perché non conoscono regimi di qualunque colore politico. Se Taiwan ha partecipato per otto anni all'Assemblea come osservatore, convivendo senza problemi con la presenza cinese, mentre oggi il Governo di Pechino pretende la sua esclusione, è evidente per noi la motivazione politica di tale esclusione

dell'Assemblea mondiale della sanità e, dunque, dell'organizzazione mondiale della sanità e affinché faccia di tutto perché Taiwan possa essere invitata ancora una volta all'Assemblea in qualità di osservatore esterno.

a divampare le fiamme, come riporta un quotidiano questa mattina. La domanda è obbligatoria: ma che rifiuti conteneva la Eco X di Pomezia se, a distanza di tredici giorni, ancora bruciano o, addirittura, si riaccendono?

Si sarebbe potuto prevedere ed evitare. Chiediamo quindi al Governo per quale motivo, all'esposto presentato nel novembre 2016 dagli abitanti della zona Castagnetta Cinque Poderi, non abbia fatto seguito l'intervento di nessuna istituzione e/o autorità preposte ai controlli ambientali. Vorremmo anche sapere se l'attività dell'azienda Eco X risultava regolarmente autorizzata all'atto dell'incidente; quali accertamenti sono stati disposti sulle ricadute al suolo degli inquinanti, con particolare riferimento alle produzioni agricole e zootecniche presenti nella vasta area interessata dalla nube tossica. Soprattutto, chiediamo attenzione sul fatto che i cittadini, nonostante le rassicurazioni da parte delle istituzioni, continuano ad accusare forti malori fisici. Nonostante il Ministro della salute abbia escluso la presenza di amianto, la Procura di Velletri ha aperto un'indagine per provare il contrario. L'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha deliberato il calendario della prima audizione di approfondimento: il prossimo 24 maggio verranno ascoltati il direttore dell'ARPA Lazio, Marco Lupo, e il procuratore della Repubblica di Velletri, Francesco Prete. È improcrastinabile, però, predisporre, di intesa con la Regione Lazio, un urgente intervento di bonifica su tutta l'area, anche al fine di prevenire l'eventuale infiltrazione al suolo e nelle falde acquifere di ulteriori carichi inquinanti. È possibile che, se è vero quanto riportato dal procuratore capo di Velletri in conferenza stampa, nel 2010 sia stata data l'autorizzazione ad operare da parte della Regione ad un impianto senza neanche la certificazione antincendio? Il sindaco di Pomezia, nel corso di un audizione in Commissione ambiente al Senato, ha affermato che nel 2015 la Regione Lazio ha rilasciato un'autorizzazione ad aumentare la quantità di rifiuti non pericolosi, ma comunque infiammabili da trattare nell'impianto. Qualcuno si è preoccupato del fatto che quell'impianto potesse operare in sicurezza? Di che tipo di rifiuti parliamo se - lo ripeto - tornano a bruciare a un passo dalle scuole di Pomezia? Infine, sia posta attenzione puntuale sul fenomeno sempre più generalizzato e frequente degli incendi ad impianti di questo tipo sul litorale sud di Roma, perché il *business* dei rifiuti è oggetto di interessi e affari da parte delle organizzazioni criminali mafiose. Concludendo, una richiesta al Ministro dell'interno. Se non è stato fatto precedentemente, si avvii un controllo accurato degli assetti societari e delle certificazioni necessarie. sono un'area vasta e una enorme comunità umana che esigono il diritto alla salute e la trasparenza assoluta negli atti e sull'informazione fornita. Occorrono controlli pubblici a 360 gradi.

una vergognosa limitazione della libertà di stampa, in una Nazione che già ha una legge sulla *governance* del servizio pubblico che ci invidiano tutte le dittature del mondo, perché è in mano al Governo la scelta del direttore e di tutti i direttori dei vari telegiornali ("PD1", "PD2", "PD3", "RainewsPD24"). Questo peraltro è un attacco che scatta adesso e, guarda caso, come dichiara Orfini, c'è qualcosa che riguarda il funzionamento della democrazia italiana e che dovrebbe allarmare tutti quanti. E infatti sono stati allarmati anni fa: ricordo che per il caso Ligresti-Cancellieri

adesso non più, perché forse era quella di De Benedetti, di Caltagirone e dei vostri amici), a Palazzo Grazioli avrebbero dovuto fare chiarezza di fronte al Paese. Ecco, se noi a queste dichiarazioni togliamo il riferimento a Palazzo Grazioli e ci mettiamo Rignano sull'Arno, forse capiamo a che punto, dove o quando il PD ha perso qualsiasi decenza nel mantenere l'informazione libera in questo Paese, senza neanche mai fare, tra l'altro, una legge sul conflitto di interessi. Ci confronteremo, mercoledì prossimo, con tutta la dirigenza RAI sull'informazione vergognosa che continua a esserci in televisione da parte del servizio pubblico e sulle dichiarazioni di questi signori, che oggi leggiamo su "Il Fatto Quotidiano", uno dei pochi giornali liberi che non appartiene a voi e che per questo attaccate quotidianamente, non solo i giornalisti, ma anche la procura. Peggio del peggior Berlusconi.